*dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro della salute:* «Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 2022, n. 2, recante disposizioni urgenti per consentire l'esercizio del diritto di voto in occasione della prossima elezione del Presidente della Repubblica»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

Signora Presidente, nel 2021 ci sono stati 1.404 morti per infortuni sul lavoro. Di questi, 695 sui luoghi di attività, con un aumento del 18 per cento rispetto al 2020. Anche questo fine settimana è stato funestato dalle morti bianche con altri tre infortuni, all'indomani della tragica fine di Lorenzo Parelli, lo studente di diciotto anni che ha perso la vita nel suo ultimo giorno di formazione.

Se ogni morte sul lavoro è una morte di troppo, quella di Lorenzo, avvenuta in un contesto che doveva essere persino più sicuro visto che coinvolgeva giovani studenti impegnati in un percorso di alternanza scuola - lavoro, è ancora più insopportabile e difficile da accettare. In Italia si è di fronte ad una strage infinita, dice testualmente «L'Osservatore Romano». Il 21 gennaio scorso, infatti, un ragazzino friulano di diciotto anni, Lorenzo Parelli, ha perso la vita in un incidente sul lavoro. Mio figlio - ha detto la madre, Elena Dentesano - è uscito per andare a scuola e non è più tornato. Un fatto straziante, inaccettabile, che ha colpito e deve far riflettere. Per la CISL, lo *stage* in un'azienda dovrebbe garantire il futuro ad un giovane, non condurlo alla morte. Per la Gilda degli insegnanti non possiamo pensare di esporre i nostri studenti allo sfruttamento, o peggio, a incidenti. Lo studente friulano è morto lavorando gratis per maturare crediti formativi. La scuola è altro. Signora Presidente, a mio giudizio questo è anche il frutto avvelenato del neoliberismo praticato da questo Governo che si avvale del pensatoio liberista Bruno Leoni, finanziato da ENI, Confindustria, Autostrade, Rai, Generali, Fastweb, Exxon Italia, British American Tobacco, Vodafone, Google, Diana Bracco e dal finanziere svizzero Tito Tettamanti, da cui il Governo pesca consulenti. Chiudo e la ringrazio, signora Presidente, con l'invito a riflettere sui nostri tempi, sulla legge n. 107 del 2015, ma soprattutto su quel feticcio denominato neoliberismo dittatoriale che, non avendo alcuna cura o rispetto per la vita umana, ha degradato le persone al rango di merci. Grazie per l'attenzione. Il Senato è convocato a domicilio. La seduta è tolta